L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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 Comunico che in data 7 novembre 2020 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno*: «Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 2020, n. 148, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020» Comunico che in data 9 novembre 2020 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze*: «Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» La Giunta per il Regolamento, riunitasi il 10 novembre 2020, ha espresso il seguente parere: «In via transitoria, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica in corso, per le audizioni delle Commissioni del Senato e delle Commissioni bicamerali per le quali trova applicazione il Regolamento del Senato, è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori, ferma restando la presenza in sede almeno del Presidente o del Vice Presidente della Commissione e del capo dell'Ufficio di segreteria».

un grande sindacalista, un grande politico del nostro Paese, a sessantatré anni dalla sua scomparsa. Costui ha dedicato tutta la vita agli altri, alla lotta per la giustizia sociale per assicurare un futuro migliore a chi non aveva nulla, ai braccianti, a chi era sfruttato, agli ultimi, a chi non poteva andare a scuola. Cominciò a lavorare nei campi a dieci anni a causa della prematura scomparsa del padre e a diciotto era già segretario del circolo giovanile socialista di Cerignola, la sua città natale. A ventuno anni divenne segretario della camera del lavoro di Minervino Murge e a ventinove, cioè nel 1921, fu eletto deputato mentre era in carcere a Lucera (era stato arrestato in seguito a un grande sciopero antifascista in Puglia). La sua elezione ebbe del clamoroso e avvenne nonostante il clima terribile di intimidazione che le squadracce avevano messo in atto a Cerignola e in tutta la Puglia, dove era molto forte la resistenza al nascente fascismo. Di lì a poco venne condannato a dodici anni dal cosiddetto tribunale speciale per la difesa dello Stato e si rifugiò prima in Francia e poi in Unione Sovietica, per poi tornare di nuovo in Francia, dove continuò la sua azione fino a che venne arrestato e poi estradato in Italia. Nel 1943 fu liberato e riprese la sua azione per la costituzione di quella che sognava potesse essere la casa comune di tutti i lavoratori, e cioè la Confederazione generale italiana del lavoro. deputato all'Assemblea costituente e poi eletto di nuovo deputato nella I e nella II legislatura. Condusse una vita davvero intensissima, senza mai risparmiarsi e indietreggiare nemmeno di un centimetro sulle sue battaglie sue battaglie per l'affermazione del valore sociale e culturale del lavoro, con salari che consentissero di far uscire definitivamente dalla povertà i braccianti e gli operai e per l'affermazione dell'indipendenza del sindacato dalla politica. Lui sognava un sindacato aperto, democratico e plurale che riunisse tutti i lavoratori senza distinzione di provenienza ideologica o di partito, perché era convinto che solo l'unità e accelerare il progresso sociale ed economico del Paese, fondato sulla Costituzione repubblicana, e l'emancipazione delle classi più deboli. In tema di unità soleva dire - lo ripeteva davvero spesso - che i lavoratori, quando si dividono, perdono. Subito dopo la guerra capì che il Paese aveva bisogno di una visione nuova e moderna e così lanciò il piano del lavoro, che aveva come unico obiettivo l'interesse comune del Paese, e coniugava le esigenze dei lavoratori e quelle degli imprenditori, dando ai primi un salario equo e, quindi, una capacità di spesa che sostenesse la domanda di prodotti e servizi e premiasse gli investimenti e lo sforzo produttivo degli imprenditori. Oggi classificheremmo le sue politiche sotto il grande cappello delle politiche espansive; le chiameremmo politiche espansive e di sostegno alla domanda interna; politiche che troveranno però applicazione anni dopo rispetto alla loro ideazione, negli anni Sessanta, e determineranno il successo produttivo del nostro Paese negli anni del cosiddetto *boom* economico. Di Vittorio era uno dei pochi grandi del sindacalismo italiano che proveniva dal movimento dei braccianti agricoli e non da quello degli operai. Ha vissuto e lottato in decenni difficilissimi, segnati dalla dittatura, dalla repressione feroce, da ben due guerre mondiali, dalla contrapposizione ideologica fortissima e poi dalla guerra fredda. ciò senza mai rinunciare ai propri principi, ai propri sogni e a ciò che riteneva un dovere imprescindibile, cioè la difesa dei deboli, degli ultimi, di chi non aveva voce. Ricordare Giuseppe Di Vittorio oggi non è solo un giusto e doveroso tributo all'uomo e alle sue battaglie per l'emancipazione della società e per i diritti dei lavoratori; non è solo una commemorazione di maniera. Quelle lotte purtroppo sono attualissime, perché le battaglie sul cottimo, sulla precarizzazione e sulla dignità del lavoro; le lotte per un salario equo che consenta una vita dignitosa e permetta di far crescere i propri figli, farli studiare e diventare protagonisti della società sono tutti temi che, purtroppo, sono riapparsi prepotentemente negli ultimi anni, gli anni della *gig economy*. *(Applausi).*

Signor Presidente, colleghe e colleghi, è un onore per me oggi ricordare Giuseppe Di Vittorio da parlamentare, da componente della Commissione lavoro del Senato, da donna dirigente sindacale che ha trascorso la vita nella CGIL. Un grande antifascista, un Padre della Patria, un politico e un grande sindacalista, Di Vittorio è stato un protagonista della nostra storia del sindacalismo mondiale, un esempio per tante donne e uomini che si sono con lui e dopo di lui battuti per i diritti e la dignità del mondo del lavoro. Di Vittorio nasce nel 1892 in un Italia liberale e agricola, in una fase di inasprimento dei conflitti sociali e territoriali, in un contesto in cui lavoratori e braccianti

Quando muore, nel 1957, lascia una Repubblica democratica fondata sul lavoro alla vigilia del *boom* economico e industriale nella quale, anche e molto grazie al suo contributo, lavoratrici e lavoratori sono riconosciuti, hanno iniziato un percorso di progressiva affermazione dei diritti hanno trovato rappresentanza politico-parlamentare e sindacale. Il racconto del suo funerale fatto da Pier Paolo Pasolini per «Vie Nuove» descrive perfettamente questa trasformazione, la capacità che Di Vittorio ha avuto di costruire una rappresentanza che è fatta di fisicità, fatica condivisa ma anche di emancipazione, di crescita personale e cambiamento organizzato. «Non ho mai visto gente così, a Roma. Mi sembra di essere in un'altra città» scrive Pasolini. «Migliaia e migliaia di uomini e di donne, quasi tutti vestiti con abiti che non sono di lavoro, ma neanche quelli buoni, della festa: gli abiti che indossano la sera, dopo essersi lavati dall'unto o dal fumo, per scendere in strada, sulla piazzetta». Dice ancora Pasolini «Incalliti dappertutto. Ma come il feretro è appena passato (...) vedo dal loro atteggiamento che qualcosa accade dentro di loro. Uno, davanti a me, piega un po' la testa da una parte: vedo la guancia lunga, nera di barba e il pomello rosso. La pelle gli si contrae, come in uno spasimo: piange, come un bambino. Guardo anche gli altri. Piangono, con una smorfia di dolore disperato. Non si curano né di nascondere né di asciugare le lacrime di cui hanno pieni gli occhi». Ecco, piangevano un uomo, un sindacalista, un *leader* che aveva dedicato a loro - ai braccianti e ai lavoratori - tutta la propria vita, aiutandoli a prendere coscienza di sé, a diventare quello che lui chiamava il popolo lavoratore, che riteneva il senso stesso dell'Italia della Repubblica, tanto che non c'era separazione, in lui, tra l'interesse dei lavoratori e l'interesse generale del Paese. Da questa convinzione profonda deriva anche il valore centrale che ha sempre riconosciuto all'unità dei lavoratori e, quindi, delle organizzazioni sindacali che li rappresentano, convinto che solo il sindacato e solo un sindacato unitario, non corporativo, mai subalterno e rispettoso della funzione delle imprese, potesse tenere insieme gli interessi dei lavoratori e creare una comunità popolare e nazionale. Non c'era nulla che non fosse disposto a sacrificare per l'unità dei lavoratori, a differenza di altri storici dirigenti comunisti. Per lui, la prima appartenenza restò sempre quella al mondo del lavoro, e così anche la condanna all'intervento sovietico del 1956 in Ungheria fu motivata proprio dall'assumere il punto di vista dei lavoratori e dalla convinzione che la democrazia fosse sempre la scelta da preferire per difenderne gli interessi. Di Vittorio aveva fiducia nei lavoratori, aveva fiducia nelle persone, aveva fiducia nella Repubblica e nella società italiana. Come ha scritto Bruno Trentin in una lettera alla sorella, anche in modo ingenuo Di Vittorio vedeva nella società capitalistica italiana la ricchezza che poteva essere prodotta, e che non lo era, piuttosto che la povertà esistente, ed era l'idea della ricchezza a entusiasmarlo. Anche il contributo che ha dato in Assemblea costituente ha permesso di affermare la rappresentanza sociale come pilastro dello Stato democratico, strumento di partecipazione dei lavoratori agli indirizzi politici nazionali, grazie a un sindacato libero, libero, democratico, indipendente, orizzontale, unitario; un modello di sindacato che ha poi fatto vivere in CGIL, cui seppe dare autonomia, identità, strategia economica, sindacale e politica, voglia di stare al passo con i tempi per restare sempre in contatto con chi lavora. In questo c'è anche una proiezione sull'organizzazione dell'esperienza personale di Di Vittorio, che non si rassegna a un destino di ignoranza. Da autodidatta riesce a diventare *leader* sindacale e politico, stimato e riconosciuto, e si convince che conoscenza e cultura sono strumenti di emancipazione, di uguaglianza, di cambiamento, e qui c'è quella capacità di ispirare, di far identificare e di guidare al meglio. Lo dice lui stesso in un discorso al II Congresso della cultura popolare a Bologna, nel 1953: nel 1953: «Io credo di essere rappresentativo di quegli strati profondi delle masse popolari più umili e più povere che aspirano alla cultura, che si sforzano di studiare e cercano di raggiungere quel grado del sapere che permette loro non solo di assicurare la propria elevazione come persone singole, di sviluppare la propria personalità, ma di conquistarsi quella condizione che conferisce alle masse popolari un senso più elevato della propria funzione sociale, della propria dignità nazionale e umana». Ecco, nel ricordare oggi una figura come Di Vittorio, non possiamo non pensare a quanto possa ancora essere d'esempio e di ispirazione per tutte e tutti noi, per le lavoratrici e i lavoratori, per le nuove generazioni. Per Per concludere, prendo in prestito le parole di Luciano Lama, che una volta spiegò nel modo seguente cosa c'è da imparare da Di Vittorio: «Il coraggio di affrontare la realtà, anche quella che non ti piace. Lo sforzo costante di non appagarsi della superficie, ma di vedere quello che c'è sotto le cose. Infine, l'abitudine a pensarci su, a non essere frettoloso nei giudizi, ma poi ad avere il coraggio di esprimerli anche controcorrente».

deputato eletto nel 1946 all'Assemblea costituente e, quindi, uno dei Padri costituenti. Leggendo la biografia di Giuseppe Di Vittorio non può sfuggire la grandezza della persona: di famiglia povera di braccianti, costretto a lavorare a partire dai dieci anni, ha avuto comunque la forza di studiare, di imparare a leggere, a scrivere, ma, giovanissimo, già a dodici anni, ha avuto l'intelligenza, la forza, la lungimiranza e - secondo me - proprio lo spirito interiore per organizzare

l'interesse per le classi più deboli, a partire dai contadini che rimanevano comunque emarginati nelle campagne, ma anche la classe operaia nelle città che si andavano a ingrandire. Ciò che mi ha sorpreso è proprio la visione, la lucidità e l'incredibile vita che ha vissuto

venne incarcerato più volte: la prima volta da ragazzo e, poi, con lo scioglimento del Parlamento e dei sindacati, venne condannato a dodici dal regime fascista. Riuscì a scappare, andò in Francia, e comunque, ogni volta che si recava in un altro Stato, riusciva a lavorare sempre per il sindacato, a favore dei lavoratori. Lo fece in Francia, in Unione Sovietica e in Spagna, lottando per la Resistenza.

Riuscì anche a tenere delle posizioni distinte da quelle del proprio partito. Egli entrò poi nel Partito Comunista, ma riuscì ad assumere delle posizioni difficili,

si distinse dalla posizione di Togliatti rispetto all'invasione delle truppe sovietiche in Ungheria per la repressione della rivolta. Egli pronunciò delle

Per una persona del suo livello, contrapporsi al segretario del proprio partito fu veramente un atto di grandissimo coraggio. A livello di

il parere ufficiale. Tuttavia, egli continuò nella sua grandissima azione di sindacalista e - ironia della sorte

quando c'è un credo tanto importante non solo per se stessi, ma anche a difesa di categorie, si può accettare di vivere incredibili pericoli e anche la carcerazione; alla fine questo lavoro paga, come si vede anche dai diritti che i lavoratori hanno per fortuna ottenuto.

ricordare oggi la figura di Di Vittorio non può avere solo un senso celebrativo. Si tratta di una grandissima figura del Novecento, che ha segnato la storia del nostro Paese, del movimento operaio e contadino e di quello straordinario processo storico per la conquista dei diritti, della giustizia sociale e della democrazia. Ricordarlo oggi potrebbe significare, per noi, avere consapevolezza dello spirito e della tenacia con cui egli affrontò quel periodo. Di Vittorio era un uomo del suo tempo, nato nel 1892: due guerre mondiali, il passaggio da un'economia fondata sull'agricoltura a un'economia industriale, un cambiamento radicale dal punto di vista sociale. Di Vittorio era preoccupato. Trentin dice che aveva un'angoscia sia come uomo, sia come CGIL, temeva di non svolgere un ruolo riconosciuto e riconoscibile sullo sviluppo della società contemporanea. In sintesi, è il significato del vero riformismo del vero riformismo e in fondo è lo stesso problema che abbiamo noi oggi, colleghi e colleghe: essere all'altezza del nostro tempo, e non per registrarne le difficoltà e le contraddizioni, ma per svolgere un ruolo capace di innovare, di cambiare, di dare senso alla politica e di combattere le disuguaglianze, di dare una funzione nazionale alla classe dirigente. Questo è quello che fece Di Vittorio. Voglio ricordare solo alcuni elementi di quella grande esperienza, fra cui il Patto di Roma del 1944. Di Vittorio, con Bruno Buozzi e Achille Grandi, dà vita all'unità sindacale. Quella fu un'ispirazione che animò tutta la vita di Di Vittorio: l'idea che l'unità del mondo del lavoro fosse la chiave fondamentale della trasformazione e della funzione nazionale del sindacato, non semplicemente rivendicativa,

per evitare che il movimento operaio e contadino si riducesse a una semplice funzione rivendicativa fine a sé stessa. Ci fu un famosissimo Ci fu un famosissimo convegno, che rappresentò una grande novità per questo Paese, organizzato dalla CGIL, sul Patto del lavoro e tutti gli economisti più importanti del nostro Paese fecero riferimento e si confrontarono con quell'impostazione. Fu un modo molto innovativo per svolgere una funzione. Pensate solo all'impegno che Di Vittorio bracciante ebbe nel contrastare le posizioni contro la meccanizzazione dell'agricoltura, che venivano esattamente anche dal sindacato, anche dalla CGIL, anche dai braccianti. Voglio anche ricordare il Congresso di Napoli del 1952, quando lanciò la proposta di uno statuto dei diritti dei lavoratori. Ci si arrivò - come sappiamo - solo nel 1970, su impulso di Gino Giugni e Giacomo Brandolini, ma certamente anche quella fu una grande intuizione. Vorrei dire, colleghe e colleghi, che noi oggi siamo di fronte allo stesso problema. Il lavoro è cambiato radicalmente: abbiamo bisogno di riscrivere le basi fondamentali dei diritti dei lavori, in questo caso, e non solo dei lavoratori. Non voglio e non posso dimenticare, poi, il 1956: la sua condanna fermissima e decisa dell'invasione da parte dell'Unione sovietica dell'Ungheria, un passaggio difficilissimo per Di Vittorio. Egli si iscrisse al Partito Comunista nel 1924. Di Vittorio, a fronte di un pronunciamento unanime della direzione del Partito Comunista Italiano, si assunse la responsabilità, in qualità di segretario generale della CGIL, di prendere una posizione netta, un giudizio complessivo sul socialismo reale e sull'idea di democrazia. Questi accenni mi servono per dire che è molto lontana dalla verità una rappresentazione di Di Vittorio solo come un capopopolo autodidatta, dall'oratoria trascinante, come una figura dalle caratteristiche neopopuliste: non è così. Di Vittorio è stato un grande riformatore: nel suo tempo ha avuto una visione avanzata, affermando un'idea di libertà di pensiero che, in una dinamica ideologica rigida e contrapposta, ha rappresentato uno straordinario contributo, una ricchezza. Se oggi si parla di autonomia del sindacato un merito grande ce l'ha certamente Di Vittorio: autonomia del sindacato, della CGIL, in rapporto, prima di tutto, con il Partito Comunista; insomma, un riformatore. Ecco cosa dobbiamo imparare noi: libertà di pensiero; anzi, prima di tutto pensiero, poi libertà di pensiero, autonomia, coraggio di vedere il cambiamento che ci riguarda e che va interpretato.

un nostro ex collega, nipote di Benedetto Croce, che sedette tra questi banchi nella X legislatura soltanto per sette giorni, essendosi poi dimesso, è autore della voce «Giuseppe Di Vittorio» nel Dizionario biografico degli italiani. Da questa voce, redatta da Piero Craveri, desidero trarre alcuni spunti per il ricordo del grande sindacalista pugliese, politico ed esponente dell'antifascismo che fu Giuseppe Di Vittorio.

«Le vicende della sua infanzia e adolescenza, riferite da lui stesso o da altri, sono già tutte cariche di significati univoci, perché precoce è la leggenda che segnerà per tutta la vita la sua figura di militante sindacale e politico, che si forma in quell'angolo di Tavoliere tra Cerignola, Canosa e Minervino Murge. Il Di Vittorio partecipò alle agitazioni della sua lega bracciantile a dieci anni. Nel 1904 durante uno sciopero generale gli morì accanto il coetaneo e amico Ambrogio, falciato dal fuoco della truppa. Nel 1907 fondò a Cerignola il Circolo giovanile socialista e l'anno seguente entrò nel direttivo della lega che aveva Antonio Mineo per capo; nel 1911 era segretario della Camera del lavoro di Minervino Murge. In questa precocissima parabola si compiva la prima formazione propriamente sindacale del Di Vittorio, i cui connotati essenziali erano la lega, lo sciopero, il contratto, l'orario e la tariffa», secondo i valori espressi dal sindacalismo bracciantile pugliese. Sarebbe anche troppo lungo voler sintetizzare i colleghi hanno ricordato alcuni tratti salienti della sua vita - la straordinaria parabola che ebbe inizio nel primo decennio del Novecento nelle campagne pugliesi: attraversò la storia d'Italia, orfana della democrazia, e i suoi momenti più critici e oscuri e si estese fino alla Francia e all'Unione Sovietica. Ebbe anche parte nella Guerra civile spagnola, fino alla nota non condivisione - ricordata poc'anzi dal collega Errani - delle posizioni ufficiali del Partito Comunista Italiano sull'invasione e sulla repressione della rivolta antisovietica in Ungheria nel 1956. Allo stesso modo il consolidamento dell'azione sindacale della stessa organizzazione con precisi obiettivi politici fu sicuramente uno dei punti fermi che costarono alla sua vita non solo talvolta interlocuzioni eterogenee contrapposte, ma anche il totale riconoscimento storico e sociale del legame tra soggettività umana e lavoro, tra mondo dell'essere e quello del fare, tra libertà e volontà, tra democrazia e diritto. A proposito di queste eterogenee interlocuzioni nel segno di creare e mantenere condizioni quanto più possibile ampie sulle questioni del sindacato e della legittimazione non esitò nel 1902 a dichiarare, nell'indipendenza che lo contraddistinse fino alla fine, non so portare la maschera della menzogna. Al mondo vivono migliaia di uomini lavorando alla giornata. Così lavorerò anche io (...)». Di Vittorio entrò nell'Assemblea costituente, portò i valori e la vita vissuta del mondo sindacale al quale apparteneva e per il quale aveva combattuto, come ho detto, già dall'età di dieci anni. Mi ha sempre particolarmente colpito durante la sua carriera politica una frase che egli proferì in risposta

fossero la zappa e la vanga, avendole usate tutte e due. Credo che sia un insegnamento fondamentale. In ultimo, Presidente, mi preme ricordare la sua vita che è stata sempre all'attenzione dell'unità sindacale, dell'unità del movimento dei lavoratori. Ho una lunga militanza nella CISL, un altro grande sindacato italiano, ma quando noi ragazzi in formazione sindacale

dei lavoratori. Penso che la sua biografia sia testimonianza per i giovani ragazzi e le giovani ragazze di oggi.

Signor Presidente, intervengo sui fatti che sono accaduti a Como

di clandestini, comunque di immigrati non in possesso di regolare permesso di soggiorno. Il più doloroso, senz'altro, è stato l'accoltellamento di don Roberto, che ha dedicato tutta la sua vita all'accoglienza degli emarginati e dei senzatetto, ai problemi appunto di questa comunità, comunque assistita da molte persone, che vive e dorme sotto un porticato. La scorsa settimana si è verificato un ulteriore gravissimo episodio. Una donna, all'ingresso di un supermercato, è stata avvicinata da uno straniero, che abbiamo scoperto non essere in possesso del permesso di soggiorno e

giusto) ha seguito questa donna e, in prossimità di un posteggio, le ha usato violenza. Ci sono dei testimoni e poi è stato arrestato, così come è stato arrestato l'omicida di don Roberto. dei cittadini comaschi, così come quella di tutto il resto d'Italia, sia una delle priorità. Non è possibile che ci siano delle persone che girano per il nostro Paese senza avere il permesso di soggiorno, senza avere un titolo un titolo e che, nonostante l'aiuto di tante persone, ritengano di delinquere e lo continuino a fare. Questo non ce lo possiamo permettere. Ogni volta che leggo che una donna violentata o molestata è un dolore per tutti. Non è possibile che le persone non possano girare per la propria città e che addirittura un atto generoso per affermare «guarda che ci sono»,

e definitivo per non vedere in giro, nelle nostre città, persone che vogliono delinquere e che, a parte tutto, non sono riconoscenti. Non è possibile rimandare sempre tutto al fatto che ci sono dei problemi psicologici o psichiatrici: non esiste. I nostri cittadini hanno diritto alla sicurezza, che deve essere la prima tra le priorità che vanno perseguite. *(Applausi)*.

caso è venuto alla ribalta qualche giorno fa e impone alla nostra coscienza più di un quesito e qualche perplessità. Possiamo starcene tranquille, quando milioni di donne sono private delle più elementari libertà, sottacendo a questa continua violazione dei diritti umani? Poiché con questi Paesi abbiamo relazioni commerciali intense e consolidate, continuiamo a far finta di niente? Possiamo continuare a conferire medaglie e onorificenze al re saudita Mohammad bin Salman che ostenta ufficialmente un impegno sociale e un profondo interesse per attività culturali e umanitaria a destra e a manca, e perciò premiarlo, quando ancora ad esempio non si è chiarito il delitto del giornalista saudita dissidente Khashoggi, consumato nell'ambasciata saudita in Turchia? Re Salman nel 2018, con astuzia e certamente con mancanza di scrupoli, ha tagliato fuori tutti gli eredi al trono, relegandoli in una prigione dorata (si tratta pur sempre di alberghi a cinque ma requisendo loro un patrimonio di più di 100 miliardi di dollari, con un colpo di Stato che ricorda molto ciò che fece nel Settecento Luigi XIV, meglio noto come il Re Sole, quando eliminò l'aristocrazia francese in un sol tratto relegandola nella dimora di Versailles. Credo che non possiamo continuare così. Tanta arroganza e prepotenza deve trovare un argine e lo deve trovare in una democrazia solida come la nostra. Il nostro Governo e l'Italia tutta devono acquisire la giusta postura nei confronti di questi tiranni che ogni tanto alzano sù la testa e fanno i forti con chi protesta civilmente e pacificamente per i diritti primari, elementari, semplicemente per i diritti umani. Ce lo impone il buon senso, ancor prima che i nostri impegni internazionali. Oggi rimane la voce sempre più flebile di una donna, Loujain, un'attivista che ha affidato la sua protesta all'estrema lotta del digiuno, relegata in carcere dopo mille mortificazioni nel corpo e nell'animo, abusata sessualmente e sottoposta ad elettroshock, elettroshock, rea di aver richiesto per lei e per migliaia di altre donne la libertà di spostarsi senza il bisogno di una scorta maschile, dopo aver ottenuto il successo di avere la libertà di guidare un'auto grazie ad una campagna di mobilitazione generale. Dunque, la comunità internazionale e il nostro Paese non possono far finta di nulla; devono pretendere l'immediata scarcerazione di Loujain e riportarla a casa, altrimenti saranno complici di una grave ingiustizia. Così come non si può far finta di non vedere la sistematica violenza perpetrata sulle donne siriane rifugiate nei campi profughi turchi, che un' assurda guerra civile costringe a vivere in totale balia degli eventi di turno.

ha confermato in modo inequivocabile quanto già emerso nei giorni scorsi e che, come senatrice sarda del MoVimento 5 Stelle, avevo già denunciato in ques'Aula il 2 settembre davanti al ministro Speranza. Queste le mie parole all'epoca: «Quest'anno, prenditori senza scrupoli hanno anteposto il diritto al divertimento e il loro profitto al diritto alla salute dei cittadini. Il risultato è stato

che è la conseguenza della malagestione da parte della giunta sardo-leghista, che durante l'estate ha consentito un «liberi tutti» a vacanzieri, residenti e imprenditori superficiali. Le scelte fatte si sono ripercosse a livello nazionale in modo drammatico. Ieri Angelo Cocciu, Capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale, ha drammaticamente ammesso davanti alle telecamere di «Report» che il centrodestra scelse di tenere aperti i locali notturni e le discoteche fino a Ferragosto, pur essendo consapevole della diffusione del contagio, e che l'avrebbe fatto per rispondere alle pressioni che arrivavano dai locali stessi, come il Billionaire, che avevano contratti stratosferici con dj importanti. Ha detto proprio così, purtroppo. Si è quindi preferito tutelare il *business* di quei locali a danno della salute collettiva.

A settembre, la Giunta ha cercato di rimediare ai suoi errori varando provvedimenti improvvisati e sbagliati, come i test obbligatori per chi arrivava sull'isola, poi impugnati dal Governo e cassati dalla magistratura. Ma c'è di più. Il presidente Solinas, l'11 agosto, avrebbe prolungato l'apertura dei locali anche sulla base di un via libera del comitato tecnico-scientifico regionale. Ebbene, questo parere nessuno sembra averlo mai letto, nonostante ripetutamente richiesto dalle opposizioni in Consiglio regionale, tanto che oggi la procura ha aperto un fascicolo per indagare la Regione Sardegna per epidemia colposa. Adesso la Giunta e tutto il centrodestra sardo devono rendere pubblico questo parere; lo devono ai cittadini sardi e a tutta l'Italia, in questi giorni alle prese con una fase molto critica della pandemia che si è diffusa in autunno su tutto il territorio nazionale anche a causa di queste scelte nefaste. Auspico pertanto un immediato chiarimento da parte del Governatore della Sardegna sulle scelte politiche fatte quest'estate in merito all'apertura delle discoteche. *(Applausi)*. Signor Presidente, porto a conoscenza dell'Assemblea un caso particolare. Non è mio costume, ma vorrei che l'Assemblea traesse insegnamento da questa esperienza devastante:

il mio vuole essere semplicemente il raccoglimento di uno spunto, incluso in un lungo *post* del padre, il dottor Maurizio Federico, responsabile del Centro nazionale per la salute globale dell'Istituto superiore di sanità: un lungo *post* su Facebook ripreso da tanti quotidiani nazionali, in cui - le garantisco, signor Presidente - non vi è mai un tono accusatorio, mai un'invettiva, ma solamente parole di plauso e di ringraziamento all'ospedale Bambino Gesù, consapevoli dell'autorevolezza e anche, in alcuni dei medici, dei tratti di umanità. In quel *post* ci sono però delle domande cui il legislatore deve dare delle risposte. Una delle domande di Maurizio Federico riguarda proprio il piano B durante un trapianto di midollo osseo. Lui purtroppo ha scoperto sulla pelle di sua figlia, una figlia adottiva, non esiste nei protocolli internazionali un piano B, per cui se il sangue del donatore si dovesse rivelare, la notte precedente il trapianto, non compatibile o non idoneo o non altamente qualitativo, purtroppo non si può fare più niente, perché non si è preventivamente preso coscienza di questo. questo. Con una petizione lanciata sul sito «change.org», che ha già raccolto 5.000 firme, sarà allora avanzata una richiesta al Ministro della salute che verrà tradotta in un'interrogazione parlamentare, affinché il Ministro della salute - che immagino sia pressato dalla maledetta pandemia e chissà quanti

con un omaggio, perché l'ematologa ha detto che non esiste un piano B, perché non succede mai. Ecco, il nostro impegno come legislatori è quello di fare in modo che quel «non succede mai» che è stato un'eccezione per Lisa

Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla luce degli ultimi tragici episodi di neonati abbandonati nei cassonetti o purtroppo a volte uccisi, come nel caso del neonato di Trapani morto con il cranio fracassato, perché gettato da una finestra del quinto piano di un palazzo, noi tutti dobbiamo riflettere su questi avvenimenti; non pronunciare solo considerazioni o parole di circostanza, ma fare atti concreti, anche con provvedimenti legislativi. Solo in questo modo possiamo aiutare le mamme in gravi difficoltà e sostenerle in situazioni così complesse e difficili. Episodi simili (sono circa 400 in un anno in Italia) avvengono in ogni realtà della nostra penisola. I tragici eventi sono legati quasi sempre a mamme in preda a crisi depressive *post partum* o sconvolte dalla paura dell'isolamento e dell'abbandono, incapaci di gestire situazioni e realtà più grandi della loro età, o ancora provocati da dinamiche familiari e sociali che stravolgono l'animo e annebbiano le menti di donne o famiglie spesso già in difficoltà. Al di là dell'importanza e del ruolo fondamentale delle associazioni per la tutela delle ragazze madri o per il supporto alle famiglie in difficoltà, volevo porre l'accento sulla necessità di offrire una possibilità concreta alle mamme e ai genitori che abbandonano il neonato, non volendolo riconoscere. Questa scelta sofferta e terribile - come detto - è motivata da svariate e complesse problematiche. I neonati sono abbandonati spesso con il cordone ombelicale ancora attaccato nei luoghi più disparati, finanche nei cassonetti, esposti al freddo e alla pioggia, con forte rischio di infezioni e di *stress* termici, capaci in alcuni casi di provocarne la morte. Ben venga l'idea di istituire dei punti di accoglienza dei neonati ubicati nelle strutture ospedaliere, che possiamo definire «culle per la vita» o «culle sociali», in cui il neonato può essere lasciato in sicurezza e in anonimato e dove può ricevere l'adeguata assistenza e le opportune cure. Queste culle, che potremmo definire le moderne ruote degli esposti, come quella precedentemente presente nell'ospedale pediatrico Santissima Annunziata di Napoli (dove io lavoro), potrebbero essere ubicate in tutti i punti nascita. A tal proposito ho presentato un disegno di legge che prevede, oltre alla collocazione delle culle, tutta una serie di iniziative di sensibilizzazione e di informazione e l'istituzione di un numero verde nazionale. Diamo una risposta concreta di aiuto alle mamme, alle famiglie in difficoltà e ai neonati, vittime innocenti, affinché questa piaga così triste scompaia. [DI

terribile che c'è negli ospedali e nelle strutture sanitarie. È una denuncia che a questo punto può servire per tutte le situazioni analoghe che si stanno probabilmente consumando in ogni angolo d'Italia. Signor Presidente, cari colleghi, io pensavo di aver visto il peggio nella mia vita professionale come giornalista, avendo assistito a disastri e

di quello che ho visto in questi giorni come semplice cittadino (perché ho avuto una sfortuna, che a questo punto diventa un'opportunità) che ha potuto, che ha potuto, per quanto poteva, mettersi a disposizione di medici e soprattutto di malati in condizioni critiche, alle prese con la morte nell'ospedale di Avezzano, credo di essere stato più utile in questi cinque giorni che in due anni di attività parlamentare. Cosa voglio dire, signor Presidente? Lo dico a lei, ma mi rivolgo al Ministro della salute e anche al Presidente del Consiglio. Nella Marsica nell'ospedale di Avezzano la situazione dei contagi è fuori controllo; non solo non si riesce a fare il trattamento, ma non si riescono neanche a fare i tamponi, perché mancano le macchine per processare e mancano i reagenti. Nell'ospedale di Avezzano si è verificata questa singolare, terribile situazione, nella quale i malati Covid stanno infettando i malati degli altri reparti, perché non si è provveduto per designati per separare le due realtà. Ci sono medici e chirurghi che escono dalle sale operatorie e sono costretti a transitare nelle zone infette. Per dire dunque alla fine che cosa? Non c'è tempo, ma mi appello al Presidente del Consiglio e al Ministro della salute, perché gettino immediatamente uno sguardo in quella struttura ospedaliera, che non solo non riesce più a fronteggiare l'emergenza, ma che è diventata un problema per se stessa, perché è diventata un centro di contagio. Ci vuole quindi immediatamente un ospedale esterno, una tensostruttura, e ci vuole personale medico e paramedico, perché la situazione è assolutamente fuori controllo. La ringrazio davvero, signor Presidente.

parlamentari che mi hanno preceduto, che hanno già tracciato la biografia di Giuseppe Di Vittorio, una biografia sicuramente fuori dall'ordinario. Da bracciante poverissimo e semianalfabeta

Cerignola, Canosa di Puglia e Minervino Murge. Di sicuro quella di Di Vittorio è stata una vita avventurosa e intensa, che spesso sfiora anche i confini del mito, senza però mai perdere di vista di vista i due valori più preziosi, entrambi concreti e solidi: il lavoro e la democrazia. Sempre schierato dalla parte dei lavoratori, dei ceti sociali più deboli, Di Vittorio ha dato un grande contributo alla ricostruzione dell'Italia nel dopoguerra. Non va dimenticato anche il suo impegno per la stesura della nostra Carta costituzionale. In questo momento di grande difficoltà e di disagio che il Paese sta vivendo, vorrei evidenziare di Di Vittorio soprattutto il senso di responsabilità nazionale, che in lui sempre è prevalso, anche nei momenti tragici della giovane Repubblica Italiana alla fine degli anni Quaranta e la sua capacità di rivolgersi a tutti, come se parlasse a ciascuno, la sua capacità di parlare al cuore della gente, quindi ai braccianti di Cerignola come agli impiegati di Roma e Milano, agli operai delle fabbriche di Torino come agli intellettuali. Un messaggio attuale il suo e, in conclusione, mi piace ricordare le sue stesse parole: «La nostra causa è veramente giusta, serve gli interessi di tutti, gli interessi dell'intera società, l'interesse dei nostri figliuoli. Quando la causa è così alta, merita di essere servita, anche a costo di enormi sacrifici Quando si ha la piena consapevolezza di servire una grande causa, una causa giusta, ognuno può dire alla propria donna, ai propri figliuoli, affermare di fronte alla società, di avere compiuto il proprio dovere».

alla sanità calabrese e un minuto dopo il nuovo commissario nel frattempo nominato. Ebbene, tutte queste notizie e questi *scoop* non hanno fatto altro se non certificare il fallimento del Governo sulla sanità in Calabria. Riporto un pensiero dei calabresi, che oramai mal sopportano tutto ciò che riguarda il commissariamento in Calabria, che è la certificazione di dodici anni di fallimenti, di dodici anni di prese in giro verso i calabresi, verso la Calabria e verso la salute stessa dei calabresi. Come Gruppo Forza Italia abbiamo presentato un'interrogazione, firmata da tutti i senatori del Gruppo, rivolta al Presidente del Consiglio e ai ministri Speranza e Boccia per farci dare delle risposte e non ci fermeremo fino a quando queste risposte non arriveranno.

«Ore e ore trascorse nella vana speranza che voi, Ministro della salute, poteste aprire un varco di luce nella mia terra martoriata, popolata da gente fiera, laboriosa nella povertà, obbediente, quasi passiva al cospetto di regole ingiuste e impari. Vi dò del voi a simboleggiare il rispetto che noi calabresi abbiamo della cultura secolare, che ci impone civiltà, che ci frena nella razionale scelta di non agire con violenza. Ma siamo ormai sepolti da ingiustizie ataviche, che subiamo senza più avere la forza di destarci. Sono calabrese da sempre e per sempre. Voglio, devo poter sedare la mia coscienza con la giustizia, che crede nella Costituzione scritta da uomini giusti. In un giorno, in un attimo, le vostre ordinanze hanno spezzato ogni sogno, ogni speranza di risollevarci. anni di commissariamento hanno costretto noi ammalati a emigrare nonostante le eccellenze mediche; dodici anni di commissariamento hanno visto depotenziare i reparti, chiudere ospedali, negare il sacrosanto diritto alla salute; costretti a file interminabili per rientrare nei pochi aventi di fatto diritto a prestazioni che per legge dovremmo avere tutti. Diritti negati sull'effimera giustificazione di "risanamento della sanità calabrese", sempre e comunque a discapito di una terra abbandonata, sedata da promesse mai concretizzate. E mentre, fieri di essere un popolo che è riuscito a tenere a bada il Covid, almeno nel primo periodo, mentre le altre Regioni potenziavano i reparti di malattie infettive, qui si riducevano i posti letto negli stessi reparti. Quando non arrivavano le mascherine non c'è stata donna, madre o nonna che non ne abbia cucite, tagliando tessuti riposti nei bauli. Ma abbiamo obbedito, pregato e abbiamo riaperto le attività di nicchia, le nostre botteghe, non certo fabbriche. E mentre siamo in zona di nuovo rossa oggi, con i nostri figli che non vedono futuro, sono arrivati i banchi a rotelle, mentre le mascherine giunte sembravano veli di carta igienica. Ma secondo quale criterio, oltre quello formalmente adottato, avete inteso non solo prorogare il commissariamento, ma addirittura potenziarlo? Perché invece non siete intervenuti direttamente potenziando gli ospedali anziché sedarci con il *bonus* biciclette? A dicembre, per Natale, se saremo di nuovo liberi, le nostre tavole non saranno imbandite. Non vogliamo *bonus*, ma presenza concreta, giusta ed equa. Vogliamo continuare a vivere con e per la dignità che ci contraddistingue; reclamiamo parità, giustizia giusta, concretezza. Ministro, andate oltre gli scarni numeri, oltre le belle parole di voler sanare la Calabria».